Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale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

il disegno di legge recante disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, che si propone di promuovere l'attività sportiva presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Durante la passata legislatura, il MoVimento 5 Stelle ha presentato diversi disegni di leggi in materia di sport, tra cui spicca in particolare l'Atto Senato 646, che detta disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, prevedendo l'istituzione della figura del docente esperto in educazione motoria e le relative classi di insegnamento. Ricordo anche l'Atto Senato 972, che reca disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport, a prima firma della senatrice Maiorino. Entrando ulteriormente nel merito tecnico del provvedimento in esame, il testo si compone di 6 articoli: il primo riconosce la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, evidenziando come l'educazione motoria e la pratica sportiva costituiscano i valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile. L'articolo 2 disciplina l'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù e prevede che la partecipazione coinvolga gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. 3 dispone che l'organizzazione dei Giochi vada coordinata da una Commissione organizzatrice nazionale. In particolare, i Giochi dovranno essere articolati in due sezioni: la prima denominata «Giovani in gioco» e la seconda «Nuovi giochi della gioventù». L'articolo 4 regola le modalità di definizione per i corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive, da stipulare attraverso protocolli annuali e pluriennali tra le istituzioni scolastiche e gli organismi sportivi, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti. L'articolo 5 pone invece l'accento sulla prevenzione, prevedendo l'istituzione di un tavolo di lavoro che coinvolgerà i rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, della società scientifica e tecnico-scientifica e delle professioni sanitarie. L'articolo 6, nel normare le disposizioni transitorie e finanziarie, dispone che l'avvio in forma sperimentale dei Giochi avvenga in occasione dell'anno scolastico 2024-2025. Ciò premesso, evidenzio che il provvedimento è stato oggetto di una cospicua attività emendativa, espletata con l'obiettivo di migliorare un testo che presentava oggettivamente alcune criticità. Ad esempio, a seguito del forte contrasto delle opposizioni, è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 2, secondo cui avrebbero dovuto partecipare ai Giochi solo gli studenti con la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva. Inutile dire che questa disposizione avrebbe ghettizzato i nostri giovani, acutizzando il *gap* tra i meritevoli e i meno meritevoli. Piuttosto, riteniamo che la pratica sportiva sia una palestra di vita e di crescita personale *(Applausi)*, che debba prescindere dal voto scolastico. Un semestre andato male non può pregiudicare ai nostri figli la possibilità di praticare l'attività fisica, che apporta benefici alla loro salute psicofisica, ma soprattutto non dimentichiamo che molte famiglie appartenenti alle fasce sociali meno abbienti non possono nemmeno permettere ai propri figli di praticare lo sport. Pertanto, la scuola potrebbe sopperire a questa criticità. Il lavoro della Commissione ha permesso di migliorare il testo licenziato dal Governo anche sotto un altro punto di vista, cioè la tutela dei soggetti fragili. Non posso che felicitarmi della modifica emendativa apportata all'articolo 2, che ha previsto per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, disciplinando anche una sezione dedicata a sport di squadra, dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme. Vorrei ringraziare a tal riguardo soprattutto la senatrice Giusy Versace, che si è spesa moltissimo per questo aspetto. Ringrazio i colleghi della maggioranza e delle opposizioni che hanno sostenuto un emendamento a mia firma che reca l'obiettivo di favorire la parità di genere, disponendo che la partecipazione ai Giochi della gioventù debba tenere conto non solo della regolare frequenza delle attività sportive promosse dagli istituti promosse dagli istituti scolastici, ma anche di un'equa rappresentanza di genere. Spiace tuttavia che sia stata bocciata un'altra mia proposta emendativa per sostenere le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro, affinché le spese sostenute per la partecipazione ai Giochi della gioventù venissero finanziate dallo Stato. Evidentemente questa maggioranza non condivide il concetto che deve (o dovrebbe) scandire ogni secondo del nostro operato politico, cioè che nessuno deve rimanere indietro. Al netto degli emendamenti approvati, che recano anche le firme dei colleghi Pirondini e Barbara Floridia, non posso non evidenziare anche l'approvazione di un importante ordine del giorno della collega Elena Sironi, che impegna il Governo a reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle scuole italiane, con l'obiettivo sia di costituire dei centri sportivi scolastici sia di creare palestre, piscine e campi da gioco. A tal proposito sarebbe opportuno, a seguito dell'accorpamento degli istituti scolastici dovuto anche alla riduzione demografica, usare gli stabili non più utilizzati per l'attività didattica per finalità ludico-sportive. Il Governo dovrebbe utilizzare i fondi del PNRR e i fondi di coesione per la valorizzazione dei beni infrastrutturali già esistenti, con particolare riferimento alla scuola primaria: da Nord a Sud, infatti, a molti studenti è di fatto negato il diritto allo sport. Evidenzio che gli impianti sportivi, i campetti e le attrezzature presenti presso moltissimi istituti scolastici risultano spesso obsoleti e abbandonati. Inoltre occorre responsabilizzare i cittadini, iniziando dalla scuola primaria, a rispettare la cosa pubblica. Sotto questo profilo il testo che stiamo esaminando ha perso la grande occasione di focalizzare l'obiettivo intorno all'edilizia scolastica fatiscente e in particolar modo sulle palestre e le strutture a disposizione delle scuole. Pertanto è necessario efficientare e ristrutturare laddove occorresse, ripensare anche in chiave *green* il nostro patrimonio scolastico. Onorevoli colleghe e colleghi, come era solito ripetere il poeta Giovenale: «*mens sana in corpore sano».* Lo sport non solo costituisce la migliore forma di prevenzione e crescita psicofisica, ma è anche disciplina, impegno, aiuta a formare la propria personalità, a socializzare e a incanalare le energie dei ragazzi per renderli dei cittadini. Memorabili a tal proposito le seguenti parole pronunciate da Nelson Mandela: lo sport lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare, di unire le persone come poche altre cose riescono a fare. Parla ai giovani una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione. Mi vengono in mente le tristi immagini di Caivano e delle tante Caivano che popolano la nostra Italia. Se solo si fosse offerto a molti giovani un modo più sano per intrattenere il proprio tempo, anche iniziando con la pratica sportiva sin dalla tenera età, probabilmente molti di loro avrebbero imboccato vie meno buie. Per questo ritengo che, oltre che incrementare il numero dei manganelli - e mi scuso per aver utilizzato questo termine, perché io penso che l'amore sia il solo mezzo attraverso il quale si veicola la conoscenza -, nei territori difficili vada prima di tutto rafforzato il numero delle scuole, delle palestre, dei luoghi di aggregazione e di vita sociale. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ciò premesso e in considerazione della forte attenzione che il MoVimento 5 Stelle da sempre rivolge alla pratica sportiva, pur ritenendo che questo testo andasse migliorato sotto diversi aspetti, annuncio, a nome della nostra formazione politica, un voto favorevole.

come primo firmatario di questo disegno di legge sull'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, desidero ringraziare, in fase di dichiarazione di voto, il Presidente della Commissione spettacolo e sport, il nostro senatore Roberto Marti, e tutti i membri della Commissione per l'impegno e la dedizione che hanno mostrato nel corso dell'esame di questo provvedimento e soprattutto per aver coinvolto in maniera determinante e direi decisiva anche il Governo, che parallelamente stava portando avanti un'iniziativa simile.

il fatto che anche maggioranza e opposizione abbiano lavorato a stretto contatto senza polemiche *(Applausi)*, ma anzi collaborando e soprattutto puntando sul fatto che stiamo parlando di un di un progetto che riguarda il tema della promozione dello sport all'interno delle scuole. È inutile ricordare l'importanza dello sport per varie ragioni, soprattutto oggi, quando si parla di dedicare una particolare attenzione al mondo dei giovani per tutto quello che sta accadendo, per le tante devianze che si notano e per i tanti impegni che sono in campo per combattere

alcuni valori fondamentali come la lealtà, l'onestà, la solidarietà, il rispetto delle regole, la disciplina,

questa iniziativa e di far sì che essa potesse davvero avvicinare i giovani anche al livello agonistico, perché lo sport sia veramente un elemento di grande unione. Tutto è finalizzato a coinvolgere i giovani nelle diverse fasi della loro crescita,

e molto importante, proprio per dare l'idea dell'integrazione che serve. C'è il coinvolgimento sia delle scuole statali sia delle scuole paritarie. Il tutto è

spesso e volentieri portano i giovani su cattive strade, soprattutto nelle zone più degradate, nei quartieri periferici e vicini alla criminalità. Tutto questo può essere d'aiuto e dare

Io credo che assuma ancora più valore quando lo associamo alla crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, dei nostri giovani, degli studenti e delle studentesse, quando ci occupiamo e preoccupiamo della loro formazione sportiva e culturale. Quando penso a quale grande funzione può svolgere lo sport nel nostro Paese, mi viene in mente, a distanza di trent'anni dal suo assassinio, quale importanza gli dava nella sua missione quotidiana don Pino Puglisi. *(Applausi)*. è stata una data importante, perché la mafia decise di ucciderlo proprio nel giorno del suo compleanno, il 15 settembre 1993. Don Pino Puglisi e, come lui, don Giuseppe Diana e tanti altri avevano capito che lo sport era uno strumento fondamentale per sottrarre i ragazzi alle grinfie della mafia. Usavano lo sport per insegnare ai ragazzi i valori genuini su cui esso si fonda, e da lì da lì nasceva l'insegnamento più grande: il rispetto delle regole e il rispetto della legalità. Don Pino Puglisi lavorò costantemente perché in quel quartiere complicato qual era il Brancaccio nascesse una polisportiva, una palestra, un luogo di aggregazione sano. Non è un caso che Cosa nostra non vedesse di buon occhio questa iniziativa: il campetto della parrocchia come punto di riferimento, come luogo dove crescere e formarsi, come spazio nel quale la mafia e il metodo mafioso non possono entrare perché incompatibili. Infatti la mafia aveva deciso che a Brancaccio, un quartiere che doveva continuare ad essere sotto il controllo e il dominio mafiosi, lo sport non dovesse trovare spazio. Don Pino Puglisi aveva capito la potenza educativa della pratica sportiva, il campetto come luogo dove stare insieme, l'etica della partecipazione, lo sport per insegnare a competere guardando sempre l'altro e l'altra come persona, come pratica per insegnare le relazioni, l'inclusione. Don Pino Puglisi ha cercato per anni di far giocare i ragazzi del quartiere. Una volta completati i lavori del campetto, la mafia prese di mira quell'impianto rendendolo oggetto di vandalismi, incendi e furti, perché la mafia tenta sempre di fare questo: distruggere ogni seme di legalità che proviamo a seminare; distruggere ogni tentativo di libertà e riscatto. I mafiosi avevano capito che il campetto, quindi lo sport, stava diventando una meravigliosa forma di educazione civica, fondamentale per lo sviluppo fisico, sociale ed emotivo dei ragazzi e delle ragazze, che con lo sport si insegnava la legalità e si formavano le personalità libere dei ragazzi e delle ragazze del quartiere. Ecco, io penso che proprio nel solco dell'insegnamento che figure come don Puglisi avevano tracciato trenta anni fa, noi oggi siamo chiamati ad investire sullo sport e sulla formazione dei nostri ragazzi e delle Credo che questo valga ancora di più nei territori complicati, nelle periferie urbane, umane e materiali; pensiamo a Caivano, ai quartieri periferici che continuano a stare al centro della cronaca nera. che noi abbiamo il dovere di intervenire e io credo che dobbiamo farlo prevenendo, agendo sulle giovani generazioni, dando loro valori sani, costruendo per loro una prospettiva di vita, lavorativa e sociale. serve infatti continuare a pensare che la legalità si ripristini con i *blitz*. È un tentativo che dura il tempo del *blitz*, ma la presenza delle Forze dell'ordine e dello Stato è sicuramente necessaria. È però altresì di fondamentale importanza l'investimento nelle scuole, nella cultura e, appunto, nello sport. Anche per questo nella discussione che abbiamo avuto in questi mesi in Commissione ci siamo battuti perché i giochi della gioventù non prevedessero ostacoli. Abbiamo infatti insistito, e ringrazio la maggioranza che su questo tema cambiato idea, perché ai giochi potessero partecipare tutti, non solo chi aveva una buona media. Questo non significa non premiare il merito, ma credere nel valore più profondo dello sport come strumento in grado di dare riscatto anche a chi conosce più difficoltà. Credo sia proprio questo il nostro compito: non lasciare indietro nessuno, accompagnare chi è più in difficoltà anche attraverso lo sport. Ecco perché penso che non avremmo svolto un buon servizio se avessimo previsto di abbandonare anche solo uno studente, prevedendo, come detto nel testo base, di escludere chi in un'età così delicata come quella scolastica potrebbe trovarsi in un momento di difficoltà. Per il resto il provvedimento su cui in questi mesi abbiamo lavorato in Commissione è un provvedimento rispetto al quale abbiamo sempre avuto un atteggiamento di condivisione e propositivo. Abbiamo sempre fatto proposte concrete, presentando diversi emendamenti che sono stati discussi, ma spesso anche accolti. Per questo devo ringraziare il presidente della Commissione, senatore Roberto Marti, che ha mostrato sempre attenzione per portarci ad un testo condiviso, condiviso, diventato così un testo di legge quasi identico a quello proposto alla Camera dal collega del Partito Democratico, onorevole Mauro Berruto. Come dicevo, l'impianto su cui questa legge si fonda ci trova sicuramente d'accordo; si parla di formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, come formazione completa dell'individuo, perché agisce nella mente e nel corpo della persona per formare personalità. Si sposa indubbiamente bene con il tentativo, che sono certa arriverà a compimento questa settimana, di inserire lo sport nel testo della nostra Costituzione come valore e principio costituzionale,

che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. È una modifica che sottolinea l'importanza dello sport dal punto di vista civile, sociale e culturale. È un'azione congiunta che mostra una particolare attenzione delle Istituzioni verso lo sport, provando a garantire strutture all'altezza di tutti, a colmare lacune che ancora oggi non permettono l'accesso alla pratica sportiva in modo paritario. Sono ancora troppi infatti i divari che caratterizzano il nostro Paese, soprattutto tra Nord e Sud. Su questo aspetto il rilancio dei Nuovi giochi della gioventù può sicuramente rappresentare un'occasione. Lo dico pensando anche alla grande funzione che lo sport svolge nei luoghi e nei territori carenti di infrastrutture e di servizi. In tali luoghi lo sport potrà costruire comunità più larghe e più forti. Dobbiamo pensare ai Nuovi giochi della gioventù, e ai Giochi della gioventù che molti di noi hanno conosciuto e a cui hanno partecipato, non solo come gare, ma come palestra di relazioni e di responsabilità. Una responsabilità sociale. Ogni ragazzo e ragazza che si avvicina allo sport, che si appassiona e si impegna, rappresenta potenzialmente un bambino sottratto al reclutamento da parte della criminalità oppure alle vecchie e nuove solitudini e fragilità. vale ancora di più in tante periferie delle nostre città. La partita da giocare e da vincere è quella che ci chiama a cogliere l'occasione e l'opportunità che ci offrono i Nuovi giochi della gioventù: lanciare messaggi concreti di speranza. Devono essere l'occasione per diffondere, sensibilizzare e condividere una serie di contenuti utili per un senso civico delle studentesse e degli studenti. La preparazione alla gara non deve essere solo tecnica ed atletica, ma deve essere affiancata ad una preparazione sociale, deve educare al rispetto della comunità, alle relazioni, alle emozioni. Avremmo voluto aprire i Giochi della gioventù anche ad altre arti, quali la musica, la poesia, il cinema, la letteratura. Non è passata la nostra linea, ma continueremo a lavorarci. Nonostante questo aspetto, riteniamo che la Commissione abbia fatto un buon lavoro e che quello che ci apprestiamo a votare sia un buon testo. Per queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico. Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di esprimere soddisfazione oggi per l'approvazione di questo disegno di legge sui Giochi della gioventù. Celebriamo, in effetti, una settimana vera e propria dello sport, perché, in contemporanea, oggi si vota definitivamente l'inserimento dello sport in Costituzione. un traguardo molto importante, per chi ama lo sport ma anche per chi vede lo sport come una visione di Governo e una disciplina importante per il Paese Noi voteremo favorevolmente e con convinzione questo disegno di legge, che segue una logica di Governo già portata avanti nella passata legislatura

con la quale si è posto alla Commissione. Tale provvedimento ha avuto un *iter* molto veloce, grazie alla collaborazione di tutti i colleghi della 7ª Commissione e al lavoro svolto in modo proficuo e veloce dal presidente

ma, consentitemi di dirlo, anche per mancanza di volontà politica. Nell'analisi dei vari colleghi, io ho sentito una disamina di quelle che sono state le motivazioni per avere i Giochi della gioventù, ma nessuna assunzione di responsabilità. Io credo, invece, che ci siano delle responsabilità politiche dei Governi precedenti, in particolare dei Governi

è chiaro che la pratica sportiva è una priorità. La testimonianza di questa visione centrale dello sport

Tutti quanti consideriamo lo sport come un'opportunità trasversale, valutandolo finalmente come un potente strumento di forza evocativa e culturale. Approfitto per ringraziare in particolare il ministro Abodi, che ha seguito sempre in Commissione i nostri lavori poi anche tutti gli altri Ministri che, con grande rispetto istituzionale, hanno lasciato l'iniziativa legislativa al Parlamento, cosa non banale e non scontata. Si intenda bene che per noi conservatori non si tratta solo di un banale ripristino di una tradizione sportiva.

di far conoscere la gioia e i vantaggi dello sport a coloro che non lo hanno ancora conosciuto. Questa è la finalità dei giochi della gioventù. Per noi del centrodestra, quando si parla di sport, è chiaro che non si parla solo di attività fisica, ma si parla anche di comunità, comunità, di inclusione, di pari opportunità e del recupero di quei luoghi dello sport che per noi sono luoghi di umanità, come è recentemente accaduto di fatto, e non solo a parole,

principalmente rivolta alla pratica agonistica, seguendo la disciplina più idonea alle inclinazioni e al talento. Concludo dicendo quello che è il cuore della nostra visione politica. Per noi investire nei giochi della gioventù e nello sport non è un costo, ma è un investimento nel nostro futuro collettivo; un investimento che porterà frutti non solo nelle medaglie vinte o nei trofei alzati, ma anche nella formazione di cittadini più consapevoli, attivi e impegnati; un investimento quindi sui giovani e sui loro talenti. Finalmente tornano i giochi della gioventù e con il centrodestra lo sport torna a essere centrale nelle politiche di governo della nostra Nazione.

Comunico che, previa intesa tra i Gruppi, la discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio,

parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Bazoli, se intende intervenire.

conciliare completezza della relazione integrativa ed essenzialità nella prospettazione all'Assemblea e, dall'altro, quello di astenersi da considerazioni squisitamente politiche e di attenersi, per contro, a considerazioni più strettamente tecnico giuridiche, sul solco del dettato costituzionale e della prassi parlamentare. Il caso che occupa oggi l'Assemblea e che è stato deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dalla Presidenza del Senato riguarda una procedura di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento al presidente senatore Maurizio Gasparri. La procedura si inserisce nell'ambito di un procedimento penale che la Giunta ha esaminato, deliberando a maggioranza nel senso della ritenuta insindacabilità. Il senatore Gasparri risulta indagato, ai sensi dell'articolo 595 del codice penale, per il reato di diffamazione con mezzo della stampa, a seguito di una querela sporta dalle signore Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, Marzullo, riferita a un *post* pubblicato nel gennaio del 2015 sull'applicazione *social* Twitter, il cui tenore letterale, per conoscenza dell'Assemblea, è il seguente: «Vanessa e Greta, sesso consenziente con i guerriglieri? E noi paghiamo! Forza Italia». Va precisato all'Assemblea che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli giunsero in Siria nel 2014 quali volontarie nell'ambito di un progetto di cooperazione finalizzato a fornire in loco aiuti medici e sanitari. Le due cooperanti furono poi rapite ad Aleppo nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2014 e liberate soltanto alcuni mesi dopo, laddove alcune fonti qualificate dell'epoca asserirono che ciò fosse avvenuto a seguito del pagamento di un riscatto da parte delle autorità dello Stato italiano. Contestualmente alla pubblicazione di questo *post* sul *social network*, si sviluppava un dibattito parlamentare in Aula, in modo particolare nella seduta assembleare del gennaio 2015. Il dibattito parlamentare fu particolarmente vivo e allo stesso prese parte anche il senatore presidente Gasparri. All'esito di tale dibattito, particolarmente acceso, ci fu anche chi giunse, per effetto di quelle dichiarazioni, rese anche *intramoenia*, a richiedere le dimissioni del presidente Gasparri. A questo punto, in tema di applicazione puntuale del dettato costituzionale, è opportuno richiamare che la giurisprudenza costante della Consulta ritiene che le dichiarazioni *extramoenia*, quindi rese al di fuori del dibattito parlamentare, siano coperte dalla prerogativa della insindacabilità, a condizione che vi sia un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare e che quindi vi sia una coincidenza contenutistica sostanziale

La Giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari ha ritenuto senza dubbio che, nel caso specifico del senatore Gasparri, il nesso funzionale sia pacifico ed evidente, atteso che - *ictu oculi* - è possibile ravvisare una esatta corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni rese. In modo particolare il dibattito parlamentare del 19 gennaio del 2015 ebbe a oggetto proprio ed esclusivamente il tema dei rischi e delle criticità legati al volontariato in zone rischiose. Sotto altro profilo, sempre in materia tecnica, bisogna comprendere se vi sia idoneità dell'intervento rispetto all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In questo soccorre la legge applicativa (l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003), che ritiene protette dal tema dell'insindacabilità tutte le attività di ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletate anche al di fuori del consesso parlamentare. In questo senso, gli interventi della Corte costituzionale, in realtà già prima della legge applicativa, ma soprattutto dopo in termini di interpretazione autentica della norma, stabilivano che andasse coperta dal tema dell'insindacabilità ogni attività, anche estranea all'aura parlamentare, manifestata in atti, anche individuali, purché costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea; questo superando il tema pregresso della tendenziale indefettibilità del collegamento tra la sede delle istituzioni, cioè il luogo in cui venivano espresse le opinioni, e la vita all'esterno delle Aule parlamentari. Quindi, non vi è stato dubbio all'interno delle elezioni e delle immunità parlamentari che le dichiarazioni rese attraverso questo strumento dal senatore Gasparri andassero ricomprese in quelle da ritenere insindacabili, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe parte dall'idea che l'articolo 68 della Costituzione sia uno strumento fondamentale per l'esercizio dell'attività parlamentare e che sia in particolare necessario per lo svolgimento di una corretta, ordinata e ricca vita democratica. I parlamentari, in linea di massima, hanno la necessità operativa, proprio per dar vita e linfa alla nostra vita democratica, di potersi esprimere con la maggior libertà e il maggior agio possibile, perché le loro dichiarazioni, soprattutto quelle rese in quest'Aula, esprimono la volontà popolare. La volontà popolare

È per questo che i nostri Costituenti, nella loro saggezza e lungimiranza, decisero di introdurre un elemento che evidentemente è di garanzia e va ad alterare i normali equilibri della vita civile civile e del dibattito tra i nostri concittadini all'esterno delle Aule parlamentari. Se un una persona utilizza espressioni offensive nei confronti di un'altra persona, la legge giustamente prevede che la persona che si è sentita offesa possa ricorrere alla giustizia per vedersi riconosciuto il torto subito ed è giusto che sia così, perché evidentemente non vogliamo che le persone si facciano giustizia da sole. Deleghiamo all'autorità giudiziaria e alla sua terzietà la valutazione della gravità delle affermazioni fatte e della loro idoneità a a ledere il prestigio della persona che è stata offesa. Questo equilibrio viene modificato dalla Costituzione, in cui al cittadino "x" o cittadino medio: se a dire qualcosa che sembra offendere la tua onorabilità è un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, purtroppo il tuo interesse a preservare la tua onorabilità deve cedere il passo alla libertà del parlamentare, perché quella libertà serve a dare linfa e vita autentica alla nostra democrazia. Quindi noi dobbiamo sempre avvicinarci con questa ottica quando discutiamo di immunità e io dico che dobbiamo farlo dando pienezza all'articolo 68 della Costituzione. Io trovo che questa eccezione alla possibilità del cittadino di difendersi da un'offesa sia giustificata, dolorosa se vogliamo, ma dovuta se vogliamo fare in modo che in quest'Aula si sia liberi di esprimere le opinioni che il popolo, eleggendoci, ci ha chiesto di esprimere. Non possiamo quindi camminare sulle uova, ma dobbiamo poter parlare. Pertanto, il nostro atteggiamento - quando discuteremo del caso successivo

Il famoso *tweet* del senatore Gasparri (quello nel quale diceva: sesso consenziente coi terroristi e noi paghiamo) dice sostanzialmente due cose. Nella sua espressione il senatore Gasparri dice due cose: da un lato, pone un tema politico relativo alla gestione degli ostaggi che la nostra Repubblica fa quando degli italiani vengono catturati all'estero e, quindi, pone un tema sulla gestione degli ostaggi, ossia se dobbiamo pagare per liberare gli italiani che siano stati sequestrati all'estero. però, ne pone anche un altro: parla di sesso consenziente, e cioè dice che le due concittadine siano andate lì per questo (al di là del pagamento, al di là del sequestro), che le due persone siano partite per la Siria perché desiderose di fare sesso consenziente con i terroristi. Quando si viene a discutere in quest'Aula di questa vicenda e la discussione viene iniziata da un intervento contrario della senatrice De Petris, il senatore Gasparri interviene, ma sostanzialmente anche nelle sue dichiarazioni dice che delle sue opinioni per quanto riguarda i riscatti, i rapimenti e il terrorismo, conserva le sue tesi che verranno discusse nei luoghi a ciò deputati e non certamente in quel momento. Pertanto, il senatore Gasparri riafferma la sua opinione politica sulla tematica del terrorismo e degli ostaggi e questa è sicuramente da considerarsi coperta dall'articolo 68 sulla vicenda sul sesso consenziente, che era stata pure sollevata dalla senatrice De Petris, il senatore Gasparri dice di scusarsi se qualcuno si è sentito offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda.

una delle cose che il senatore Gasparri ha detto alla Giunta: io ho soltanto ritwittato qualcosa che era stato detto da altri, ma è evidente che il *retweet* fatto da un personaggio pubblico ovviamente attribuisce a quel messaggio una visibilità che altrimenti non avrebbe avuto. Pertanto, questo aspetto lo terrei completamente al di fuori. Dal nostro punto di vista certamente dobbiamo avere un occhio

noi consideriamo che la parte relativa alla gestione del terrorismo, ostaggi e quant'altro sia sicuramente parte dell'attività politica anche svolta in quest'Aula dal senatore Gasparri e sia chiaramente insindacabile. Riteniamo invece che la condotta, l'accusa e l'affermazione che le due concittadine fossero andate lì per fare del sesso consenziente costituiscano un fatto diverso, distinto e separato

pendente nei confronti del senatore Gasparri, sulla quale la Giunta si è espressa scudando lo stesso in quanto le opinioni espresse ricadrebbero nell'articolo 68 della Costituzione quale opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni.

Con la relazione della Giunta affrontiamo la materia del fantadiritto. Da avvocato ho studiato diritto penale, amministrativo e civile, ma devo candidamente ammettere che nel mio corso non ho mai studiato il fantadiritto, non era ancora materia di esame, nemmeno complementare. Nella relazione si citano le ormai solite, notissime sentenze della Corte costituzionale e si ripete sempre l'assunto che, a prescindere dal tenore delle dichiarazioni *intramoenia* rese, le stesse siano sufficienti a scudare la condotta grazie al nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza tra le opinioni espresse all'esterno e quello espresso nell'ambito delle attività parlamentari. Ricordo a me stessa che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno in più occasioni delineato l'esatto ambito di operatività del precetto costituzionale, evidenziando in particolare la necessaria sussistenza di un nesso funzionale tra la condotta che si assume essere delittuosa e le specifiche iniziative ed attività parlamentari, le quali non dovranno essere ascrivibili a questioni che siano meramente politiche.

ma necessiterebbe di un raccordo con le specifiche iniziative di attività parlamentari. Ma vi è di più: occorre anche citare la sentenza della Cassazione (sempre per chi è interessato, la n. 32862 del 2019), laddove richiede, ai fini di una eventuale pronuncia di insindacabilità, un legame fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima. A questo punto, analizziamo i fatti

Questo è il *post* pubblicato su Twitter il 18 gennaio 2015. Verifichiamo quindi la corrispondenza contenutistica sostanziale con l'intervento reso in corso di seduta dell'Assemblea del 19 gennaio 2015. Intanto, c'è da sottolineare che è la senatrice De Petris a sollevare la questione, stigmatizzando il *post* proprio in quell'occasione in Aula. Dopodiché, presero la parola altri cinque senatori e poi replicava il senatore Gasparri, all'epoca vice Presidente del Senato, il quale testualmente afferma: «Signora Presidente, ovviamente non concordo con la proposta della senatrice De Petris, mentre apprezzo l'invito alla prudenza del senatore Zanda, che penso debba riguardare sia l'uso dei *social network*, sia le azioni del volontariato in territori rischiosi. rischiosi. Ovviamente, se qualcuno si è offeso del fatto che sia stata rigirata una domanda (...), perché di questo si è trattato, mi scuso con chi si è ritenuto offeso. Per Per quanto riguarda i riscatti, i rapimenti e il terrorismo, conservo le mie tesi che discuteremo nei luoghi a ciò deputati, e non certamente in questo momento». Spiegatemi come può un intervento del genere essere sufficiente al fine di far scattare le guarentigie di cui all'articolo 68 della Costituzione. L'unica cosa che emerge *ictu oculi* è - come scritto nella relazione della Giunta - non la corrispondenza tra atto *intra* ed *extramoenia*, bensì le scuse postume che il senatore Gasparri è stato costretto a fare in relazione alla richiesta di dimissioni formulata dalla senatrice De Petris, nonché l'invito a discutere le questioni nel luogo a ciò deputato. All'epoca, infatti, anche il senatore Gasparri non considerava un luogo adatto alla discussione l'Aula del Senato. Immagino invece si riferisse proprio a un'aula di tribunale. Ebbene, siamo d'accordo con il senatore Gasparri: ne discuta in tribunale e dia seguito a un sacrosanto procedimento. Sorprende, ma fino a un certo punto, anche la tempistica dell'esame di tale provvedimento. Tale atto fu deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 18 luglio 2018. l'esame non fu concluso nella scorsa legislatura? Perché è stato messo all'ordine del giorno solo ora che il centrodestra detiene la maggioranza? Chi era il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nella scorsa legislatura? Come direbbero i francesi, *ça va sans dire.* C'è da fare una valutazione generale sul ruolo che il Regolamento del Senato impone alla Giunta. Essa si colloca nel novero degli organismi paragiurisdizionali, imponendo che le decisioni prese debbono essere basate su precisi presupposti di fatto e di diritto, come accade nell'applicazione di qualsiasi istituto giuridico. Purtroppo, questo organismo sta assurgendo a un organo assolutamente politico, anzi direi politico per eccellenza, che prende decisioni fondate su presupposti corporativisti piuttosto che su un'attenta lettura delle carte. delle carte. *(Applausi)*. Cosa dobbiamo aspettarci noi da questa maggioranza? Ricordiamo con orrore la votazione del 5 aprile 2011, quando 232 deputati dell'allora PdL votarono che Ruby la notte del 27 maggio 2010 era per lo Stato italiano la nipote di Mubarak. Chissà se l'ha votato anche il senatore Gasparri. Per queste ragioni, Per queste ragioni, dichiaro il voto contrario alla relazione della Giunta.

e che aprono una discussione e una riflessione sui rapporti stessi fra l'espressione di un diritto di critica, l'espressione di un'opinione e l'attività politica in sé.

la legge n. 140 del 2003 ritiene che l'articolo 68 copra non solo le dichiarazioni rese in Aula, ma anche la presentazione dei disegni di legge, degli emendamenti e degli ordini del giorno, qualsiasi espressione di voto e ogni altro atto parlamentare, ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare. Quindi l'attività che viene resa *extra moenia* e l'attività che viene resa *intra moenia*, se dovessimo anche anche tenere conto del mutamento dei tempi, non possono essere così rigorose e matematiche. Bisogna tenere conto che, da quando è stata scritta la Costituzione ad oggi, l'attività del parlamentare è anche mutata in sé. in sé. Se potevamo pensare che l'onorevole Aldo Moro si esprimesse e facesse politica all'interno dell'Aula attraverso i suoi interventi articolati, oggi vediamo invece un'attività politica che non si esaurisce nell'attività in Assemblea o in Commissione, ma che molto viene estrinsecata all'esterno.

Dobbiamo anche ricordare che, nel corso dell'esame dei vari casi in Giunta, sono emerse delle lacune nella stessa normativa oggi prevista. Ci siamo posti anche il tema dell'espressione di un'opinione, che magari poi viene censurata a titolo di diffamazione, anche da membri del Governo che non ricoprono

Questo potrebbe e dovrebbe portare - a mio avviso - a una sorta di ampliamento delle ipotesi, proprio per adeguarsi a questo cambiamento di *mores*; *mores* nel senso che oggi la critica politica non si esaurisce magari in forbiti interventi, ma spesso ha anche delle espressioni magari più aspre

trattandosi comunque di tematica politica ampiamente discussa e appartenente di certo alla proprietà e alle argomentazioni portate avanti dal senatore Gasparri.

giuridico, le considerazioni sono anche condivisibili. È stata fatta una panoramica con la quale si è sottolineato come le espressioni e le opinioni espresse fuori da quest'Aula, che possono avere anche contenuto diffamatorio, siamo coperte dalla guarentigia *ex* articolo 68 laddove vi siano atti tipici, come interrogazioni o interventi in che riportano quasi integralmente o pressoché integralmente il contenuto delle dichiarazioni espresse fuori da essa. Ciò corrisponde alla necessità di difendere la libertà dei singoli parlamentari che devono poter esprimere ogni critica politica senza il rischio di incorrere in procedimenti anche di diffamazione a loro carico. È un principio condivisibile che è stato anche enunciato in maniera molto chiara dal collega Scalfarotto. Noi condividiamo la necessità di difendere con grande attenzione questa prerogativa, questa caratteristica legata alla funzione parlamentare e delineata in maniera molto chiara dall'articolo 68 della Costituzione.

però dimenticata di riferire che questo criterio di valutazione, anche delle parole che vengono dette dai parlamentari, si applica alla battaglia politica, cioè alla critica politica che riguarda

spesso anche di termini e di epiteti che fuori sarebbero consigliato offensivi, ma che dentro l'agone della politica non è giusto vengano considerati tali. Qui, però, stiamo parlando di una cosa diversa, perché stiamo parlando di espressioni, proferite da un esponente politico autorevole e noto, nei confronti di privati cittadini.

di una frase, scritta su Twitter, che dice: "*Vanessa e Greta**, *sesso** consenziente con i guerriglieri? **E noi paghiamo!".** Queste sono le parole pronunciate e scritte su Twitter. La chiara attitudine offensiva di tali parole non può essere scriminata neanche da un intervento in Aula del giorno successivo, nel quale il senatore Gasparri si è scusato. Esse non costituiscono una critica politica e dunque non appartengono al novero della critica politica coperta dall'articolo 68. Queste sono le ragioni per le quali noi, pur apprezzando la veste giuridica e la costruzione giuridica data dal relatore alla vicenda, non possiamo condividerne le conclusioni.

senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

parlamentari ha proposto, a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dall'onorevole Nicola Morra, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Bazoli, se intende intervenire. intervengo per dare conto delle valutazioni che ha fatto la Giunta, ricordando che questo procedimento è originato da una vicenda nella quale l'onorevole Morra è stato citato in giudizio da una società cooperativa, la "Malgrado Tutto srl", in relazione ad alcune affermazioni da lui proferite nel corso della trasmissione televisiva "L'Arena", in onda su Rai 1 il 10 aprile 2016, ritenute dalla società diffamatorie e lesive della propria immagine. In particolare l'onorevole Morra in quel programma televisivo, senatore Bazoli. Colleghi, davvero vi prego di ridurre il brusio e di non voltare le spalle alla Presidenza. Si può anche uscire dall'Aula, se non si vuole partecipare al dibattito. BAZOLI, Dicevo che in quella trasmissione, dopo aver sostenuto di dover riportare un episodio relativo alla sua visita presso il centro di accoglienza, che lo lasciava molto turbato, avrebbe sostanzialmente dichiarato di aver visto personalmente alcuni ragazzi del centro che lavoravano ai pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura senza alcuna protezione, in violazione delle norme sulla sicurezza. Riferendosi appunto a quel centro di identificazione ed espulsione gestito da quella società cooperativa e al suo rappresentante legale, si domandava «come questa persona possa gestire, e non da oggi ma da parecchi anni, soldi pubblici ma soprattutto vite umane con così grande leggerezza». Proseguiva il senatore Morra dicendo: «Io ricordo che il C.I.E. in questione o C.T.P. o quello che è stato ha anche avuto la tragica esperienza di vantare 5 suicidi e sempre con la Malgrado Tutto che gestiva la struttura». Secondo la società cooperativa queste affermazioni avrebbero riportato circostanze prive di fondamento e attribuito alla stessa fatti mai realmente accaduti e rivestirebbero quindi un carattere diffamatorio. Anche in questo caso - come in tutti i casi che ci occupano quando si parla di insindacabilità - occorre valutare non solo ovviamente l'attitudine diffamatoria delle dichiarazioni, ma anche se vi siano attività *intramoenia*, cioè attività svolte dal parlamentare all'interno

presunta o ipotetica attitudine diffamatoria, dalle considerazioni svolte in quest'Aula. Ora, nel caso di specie risulta ed è appunto emerso nell'istruttoria che abbiamo fatto in Giunta che, se è vero che le parole esatte pronunciate nel corso della trasmissione televisiva non furono oggetto di contenuto di atti tipici del senatore Morra all'interno di quest'Aula, è però vero la questione inerente alla gestione dei migranti e alla condizione dei migranti ospiti nei centri di prima accoglienza è stata al centro dell'attività politica svolta anche in quest'Aula dal senatore Morra nel corso degli anni in cui ha ricoperto la carica di senatore. Ci sono infatti numerose interrogazioni parlamentari che portano la sua firma in cui si pone all'attenzione tale problematica,

in modo che l'Assemblea ne sia consapevole, ma il dettaglio è contenuto nella relazione - le interrogazioni delle quali il senatore Morra fu firmatario o cofirmatario, nelle quali esattamente la condizione dei migranti veniva messa al centro dell'attenzione: l'interrogazione a risposta scritta del 25 giugno 2015, l'interrogazione a risposta orale del 23 settembre 2015, l'interrogazione a risposta scritta del 19 novembre 2015, l'interrogazione a risposta scritta del 22 novembre 2013, l'interrogazione a risposta scritta del 10 marzo 2015, e altri atti di cui fu cofirmatario il senatore Morra, tra cui mozioni per esempio una mozione del 13 giugno 2013 - e altre interrogazioni che riguardavano non tanto la condizione dei migranti, quanto l'immigrazione clandestina, le politiche migratorie questioni attinenti in larga misura alla condizione dei migranti. Anche sotto il profilo della contestualità delle frasi pronunciate in quella trasmissione televisiva con gli atti tipici depositati dal senatore Morra, abbiamo dovuto constatare che c'è una pertinenza, una coerenza temporale. Anche sotto questo profilo,

e, in particolare, della circostanza che sia fuori discussione che il tema dell'adeguatezza e della legalità del sistema di accoglienza fosse al centro dell'attività politica e parlamentare del senatore Morra, come documentato dai plurimi atti di natura squisitamente parlamentare depositati e dalle numerose visite ispettive effettuate nei centri di accoglienza, si ritiene corretto concludere che anche le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, sia pure non esattamente coincidenti a livello terminologico e testuale con gli atti menzionati, debbano essere ricomprese nell'ambito della insindacabilità coperta dall'articolo 68 della Costituzione, pena - ad avviso della Giunta, che ha concluso in maniera quasi unanime - una irragionevole limitazione della guarentigia che assicura la piena libertà di mandato al parlamentare, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Consulta per la configurabilità della insindacabilità. Per questi motivi la Giunta delle sia pure a maggioranza, all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dell'onorevole Morra, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

della giurisprudenza costituzionale, ma non dobbiamo neanche cadere in una sorta di meccanicismo per cui, per poter applicare l'articolo 68, dobbiamo proprio individuare una perfetta coincidenza delle parole utilizzate. Se un parlamentare, come il senatore Morra, si è occupato durante il suo mandato in particolare di quella di quella materia e se n'è occupato in molti modi e molte sedi, qui in Parlamento e nella sua attività politica fuori, e viene querelato per qualcosa che ha a che fare, se non con un'applicazione meccanica dell'individuazione delle parole, certamente con la sua attività parlamentare, pensare di poter sindacare dal punto di vista giurisdizionale quel contenuto oggettivamente politico, condivisibile o meno, ma certamente parte delle sue opinioni e delle sue attività dentro e fuori dall'Aula. Credo che in quel caso sia fuori discussione che l'articolo 68 vada applicato. Di conseguenza, voteremo a favore della relazione. Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione riconoscerà con il proprio voto in Aula la proposta pervenuta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Apprezziamo le argomentazioni logico-giuridiche che supportano l'insindacabilità *ex* articolo 68, 68, primo comma, della Costituzione in riferimento alle affermazioni espresse dal senatore Nicola Morra. Il carattere di conseguenza logico-temporale tra gli atti parlamentari presentati dall'allora senatore e l'intervento televisivo oggetto di contestazione palesano la sussistenza del cosiddetto elemento temporale fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna del parlamentare: un requisito giuridico, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che supporta quello della rispondenza contenutistica, appunto, tra atto *intramoenia* ed *extramoenia*. Il tema dell'adeguatezza e della legalità del sistema di accoglienza era al centro delle attività del senatore Morra e non solo del collega ovviamente: le numerose visite ai siti di accoglienza e gli atti ispettivi da lui presentati non recano dubbio alcuno circa la possibilità di vedere operante la garanzia di cui all'articolo 68; di più ed anche, come nel caso che ci interessa, a fronte di una non esatta rispondenza terminologica tra le parole utilizzate nell'ambito del contesto televisivo e quelle oggetto degli atti parlamentari, essendo il tutto, come evidenza, il frutto di un'azione politica unitaria alla quale non possiamo disconoscere la copertura costituzionale dell'articolo 68.

senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

questo è stata, una corsa a perdifiato - che Cesare Martinetti gli ha dedicato questa mattina su «La Stampa». Le origini, nella *epochè* tra la sua Torino e la radice nella Calabria (a Cetraro), la formazione e l'impegno cattolico, la scelta della filosofia, il magistero di Pareyson, la Germania con Gadamer e Löwith (tremano i polsi solo a pronunciarli questi nomi), l'amicizia con Eco, la RAI, la vita accademica, l'estetica, il pensiero debole - certo -, la dimensione politica (controversa, erratica), il rovello della vita personale, la montagna, il *coming out* come si direbbe oggi, gli anni del fuori, i lutti terribili; le polemiche, anche quelle sbagliate, sbagliatissime; i dissidi direbbe il suo Lyotard. Ieri la morte con quell'ironico «Ei fu» sulla sua pagina Facebook. «Ero debole», che eleganza fino alla fine, quell'imperfetto. Oggi ci consoliamo con la lezione del pluralismo e del disincanto, del dialogo, l'ermeneutica come vaccino contro gli *ipse dixit;* non è un caso che al suo Heidegger si attribuisca proprio sull'ermeneutica una smorfia sprezzante (roba da Gadamer) come strumento di falsificazione delle verità solide, ma anche come gioiosa *ars combinatoria* che restituisce e anticipa uno spirito del tempo che - celiava Vattimo - non è lo spirito santo. Tuttavia la filosofia è sempre stata e rimasta per lui domanda radicale e *thaumazein* (altro che debolismo). Ha recuperato l'innominabile Nietzsche, lo ha reso ospitale, lui così forastico per le nostre anime belle, soprattutto a sinistra. La ricezione italiana e non solo del pensiero heideggeriano gli deve moltissimo; chi non ha computato avido il suo arancione e Heidegger è con Wittgenstein il Novecento. L'ermeneutica in Italia gli deve semplicemente tutto: verità e metodo - mi perdonerà Emilio Betti, buonanima. Tormentato, tragico, divertente, religioso, impunito come diciamo a Roma; aveva uno sconsiderato bisogno di amore, come se

io prima di nascere non sapevo che il mondo fosse così interessante, dopo la morte chissà cosa trovo. Ci dirà, professore caro. A chi resta basti per ora quello che ha cercato. La ringrazio.

però io desidero anche ricordare un uomo che è stato estremamente coraggioso, una persona che ha vissuto la sua omosessualità pubblicamente in un Paese, il nostro, in cui essere sé stessi non è facile, soprattutto per persone della generazione di Vattimo che ovviamente hanno avuto da aprire porte che loro stessi hanno aperto e di cui noi più giovani generazioni ci siamo sicuramente serviti. È un uomo che si è esposto, che ha deciso di vivere in piena libertà ciò che era, di vivere le sue relazioni sentimentali, ciò che lui considerava famiglia. E credo che grazie anche ad esempi come quelli di persone come Gianni Vattimo oggi la comunità LGBT in Italia abbia diritti che sono nati anche dal loro lavoro e dal loro coraggio. Vattimo riconobbe

quindi unirmi a questo ricordo a nome di tutta la comunità LGBT italiana proprio per ricordare insieme a Gianni Vattimo una generazione di uomini e donne coraggiosi che in un Paese difficile come il nostro hanno deciso di esporsi, di vivere sé stessi in piena libertà e dignità facendo in questo modo crescere la coscienza civile di un intero Paese.